finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

grande sportivo italiano, più volte detentore del record mondiale di immersione in apnea e componente di questa Assemblea nella XII legislatura. Nato a Siracusa il 21 giugno del 1931, Enzo Maiorca è fin da giovanissimo attratto dall'amore per il mare e dallo spirito di esplorazione dei fondali marini. Nell'estate del 1956, suggestionato dal record di profondità conseguito da due pescatori subacquei - Ennio Falco e Alberto Novelli - decide di cimentarsi nella pratica sportiva delle immersioni in apnea. Soltanto pochi anni dopo, nel 1960, tocca il record di discesa fino a 45 metri di profondità, battendo il brasiliano Amerigo Santarelli, detentore del primato mondiale. È l'inizio di una grande era che vede Maiorca migliorare più volte quel traguardo, fino al 1988, anno in cui abbandonò la pratica delle immersioni, dopo aver conseguito il suo ultimo record di 101 metri di profondità. Nel 1994 viene eletto senatore nelle liste di Alleanza Nazionale ed entra a far parte della Commissione difesa. Da parlamentare si impegna in modo particolare per iniziative legislative volte al contrasto alla delinquenza minorile, alla disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali, all'istituzione del Ministero del mare, nonché - da relatore - per la conversione di decreti-legge relativi allo svolgimento di missioni internazionali di pace. Con Enzo Maiorca scompare quindi un grande sportivo, ma anche un uomo che, con generosità e spirito civico, ha utilizzato la propria popolarità per divulgare presso l'opinione pubblica l'amore per lo sport e per la natura, oltre che l'importanza della tutela dell'ecosistema e del patrimonio marino. Nel formulare la sentita partecipazione del Senato della Repubblica al dolore dei familiari, degli amici e della comunità siracusana per la scomparsa di Enzo Maiorca, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

troppo poco rispetto a quello che lui ha compiuto e, probabilmente, non sarei riuscito a restituire ai colleghi e all'Assemblea

la competizione che, in maniera superficiale, è stata percepita da tanti che lo hanno seguito nelle battaglie prima con Santarelli e, poi, con Mayol. Sono stati due i principi che hanno informato la vita di questo uomo: uno è stato quello della sfida con se stesso, poiché lui non sfidava Santarelli e non sfidava Mayol, ma se stesso;

Nel 1931 nasce a Siracusa in un paesino, in una frazione molto vicina al mare: poteva guardarlo da 70-100 metri. Questo bambino guardava l'immensità del mare, con i suoi colori, la sua rabbia, la sua forza; allora, nessuno conosceva gli abissi, nessuno sapeva cosa c'era sotto. Il bambino aveva semplicemente ricevuto dai pescatori l'immagine dei mostri marini e di quello che poteva accadere dentro e sotto quello che si vedeva, e iniziò a percepire il mare sia in misura orizzontale - come quasi tutti noi lo percepiamo - sia in una dimensione verticale, nella dimensione cioè di quello che c'è sotto.

dal guardare sott'acqua attraverso gli occhi nudi, in maniera confusa, al guardare attraverso un vetro e ad avere una percezione molto più distinta e vera di quello che sta sotto il mare, in quel mare verticale. Cosa sono gli abissi per lui lo dirò dopo. Il presidente Grasso ha citato due record importanti di Maiorca. Uno nasce quasi per caso:

ha realizzato film bellissimi, si sia lasciato trasportare nel suo film «Le Grand Bleu» in quella pessima rappresentazione di un dualismo stupido e anche un po' bizzarro e surreale tra Mayol e Maiorca, che si vedevano ogni tanto,

non era un ragazzino; quindi era l'ennesima sfida con se stesso. Poi è stato senatore, come ha ricordato il presidente Grasso, nel 1994 nel 1994 con il Governo Berlusconi, nelle file di AN; lo abbiamo ricordato con Altero Matteoli che credo sia stato il suo Capogruppo di quegli anni. Ho due ricordi che vi voglio restituire. Uno è di quando ero piccolo e l'ho conosciuto per la prima volta e, il secondo, di quando eravamo a tavola al matrimonio di un nostro parente.

a quello che la Sicilia e l'Italia avrebbero potuto essere e che in realtà non riuscivano a essere perché i siciliani e gli italiani non sapevano ben scegliere i politici e perché la macchina

Mi ricordo questa cena. Il secondo ricordo è il seguente: la prima volta che lo vidi ero a casa di una nostra parente; entrai, molto piccolo, mano nella mano con mia mamma, e non chiesi a mia madre chi fosse Enzo Maiorca,

Quel luogo era Ortigia, quel luogo era Siracusa, quello era il mare. Il senatore Alicata, con il quale ieri ci siamo confrontati, mi ha detto una cosa molto bella. Quando si è incontrato con lui - l'uno senatore e l'altro futuro senatore - ha cercato per tutto il colloquio di dargli del lei e poi, alla fine, Enzo Maiorca gli ha detto: «Ti prego, dammi del tu», e così fu. avesse nei confronti di Enzo Maiorca un grande rispetto, nutrito verso una persona che aveva raggiunto una serie di obiettivi. Gli abissi sono una cosa a parte per chi li ha praticati. quando si scende oltre i 50, 60, 70, 80 metri - e chi vi parla questa cosa l'ha fatta - non si ha la percezione tattile, si perde l'udito, perché alterato dall'acqua, e non sia ha né l'olfatto, né il gusto. Si ha solamente il contatto forte con la vita, con il respiro che si ha dentro i polmoni, e il cervello è perfettamente collegato con il singolo battito cardiaco che ti tiene in vita.

E quando ritorni verso la superficie, verso la vita e verso i colori - perché quando si è oltre i 60-70 metri si vede tutto blu - è un'esplosione di gioia, che solo chi ha fatto queste cose può percepire. Ecco perché Enzo Maiorca affermava che quando poteva andava sott'acqua non perché andava nel mare, ma andava sott'acqua perché trovava se stesso. Su questo vi voglio dire una cosa, che riguarda noi tutti. Vedete, molte volte qui, in superficie, quando percepiamo il mare orizzontale e non il mare verticale, quando non abbiamo una netta percezione di noi stessi e di quello che dobbiamo fare, quando non capiamo qual è la sfida della nostra vita, ci perdiamo. Forse in questo momento, la morale di questa vita celebrata - di questo ringrazio il presidente Grasso e i colleghi, che hanno consentito questa commemorazione stamattina - ci deve fare in qualche misura anche ritrovare noi stessi. Ritrovare noi stessi, il perché facciamo le cose e qual è l'obiettivo che dobbiamo avere, prima conoscendo e rivalutando noi stessi e, alla fine, diventando parte di un tutto. Quando a Enzo Maiorca Quando a Enzo Maiorca veniva fatta la domanda «ma tu chi sei?», lui rispondeva che era una goccia. Era la goccia di quel mare che era il tutto, di cui lui si sentiva parte. Vi ringrazio di avermi concesso di parlare stamattina, ringrazio il presidente Matteoli e il senatore Alicata, che avrebbero voluto parlare di Vincenzo Maiorca, perché lo hanno conosciuto direttamente (uno come Capogruppo e l'altro per una frequentazione nella città di Siracusa) e vi porto i saluti della moglie Maria,

per la verità poco ci sarebbe da aggiungere. Ma non posso sottrarmi dall'evidenziare le doti umane di questo grandissimo personaggio, di questo sportivo straordinario, di questo siciliano straordinario e orgoglioso e di questo grande, grandissimo italiano. italiano. Queste prove estreme le ha volute confrontandosi con se stesso e mai rivolgendosi contro i suoi temibili *competitor*, ma sempre con quello spirito di rispetto delle istituzioni, dello sport, degli avversari e della comunità. Il suo amore per la nostra Italia e per la sua Sicilia è stato straordinario; un esempio per me e per noi sportivi di straordinario valore, un qualcosa che deve rimanere non solo per tutti coloro che sono amanti del mare, ma per noi tutti italiani, che nelle prove estreme, nei momenti di grande e di assoluta difficoltà, signor Presidente, troviamo quella forza interiore che viene dalla nostra storia.

Grazie premetto che nessuno meglio di Maiorca può raccontare Maiorca e, in questo senso, voglio ringraziare il grande atleta per averci narrato con grande poesia le sue gesta. le sue gesta. Tuttavia, ho comunque cercato di cogliere alcuni aspetti della sua persona e della sua personalità, che hanno contraddistinto la sua unicità e ci hanno ci hanno consegnato una grande eredità da trasmettere. Per questo motivo, è davvero con grande emozione che ricordo oggi Enzo Maiorca - il signore degli abissi, come lo chiamarono - per aver fatto della ricerca della profondità una sua ragione di vita.

chi lo ha conosciuto di persona e chi ne conosce il mito soltanto per vie indirette, vorrei cogliere questo momento per farmi interprete e magari anche amplificatore delle gesta, dei messaggi e dei valori che Enzo Maiorca ci ha lasciato in eredità. Tanti di noi quest'anno hanno seguito le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Abbiamo gioito, orgogliosi per medaglie e vittorie, e abbiamo partecipato alla rabbia e alla delusione di chi non ha coronato i propri sogni.

dicevo, una volta spenta la fiamma olimpica, succede però sempre la stessa cosa: passati alcuni mesi, nessuno si ricorda più degli eroi nazionali. È vero, Enzo Maiorca non è stato un atleta olimpico, ma ho voluto accostarlo a quell'ambito dello sport che, forse, insieme al calcio, muove più di ogni altro le emozioni degli spettatori, per rilevare la grande caratura del protagonista che oggi ricordiamo come uno dei grandi, grandissimi miti dello sport italiano, nonostante l'immersione in apnea non sia esattamente uno sport di massa o di incassi, o comunque ispirato a qualsiasi criterio che scateni l'attenzione del grande pubblico. Cosa è, dunque, che fa diventare un grande atleta un mito dello sport, un titolare della storia sportiva scritta con la «s» maiuscola? Se ripercorriamo le varie tappe del percorso di Enzo Maiorca, possiamo captare davvero molti ingredienti di questa ricetta che possiamo chiamare vincente. Il primo ingrediente, antico quanto moderno, per questa leggenda è ciò che chiamo la storia nella storia, perché ciò che resta non sono solo le imprese e i record di Maiorca, ma anche la grande rivalità e l'agonismo con un altro protagonista di apnea, prima descritto benissimo dai descritto benissimo dai colleghi, Jacques Mayol, il quale ha fornito la stoffa per epiche narrazioni che si sono impresse nella memoria collettiva. Preparando questo intervento, mi sono imbattuta in un'intervista rilasciata da Maiorca cinque anni fa a La Spezia, uno dei luoghi dei suoi record, nell'ambito della Festa della Marineria, in cui gli fu chiesto se, nell'arco della sua carriera, durante le sue discese si sia sentito come un esploratore oppure se ogni discesa sia stata più una discesa per se stesso. Maiorca ha risposto: «No, non mi sono mai sentito un esploratore, ho sempre cercato invece di aggiungere tasselli alla mia conoscenza, alla conoscenza che ho di me», rivelandoci con queste parole le sue profonde motivazioni nel fare lo sport. Maiorca non cercava il risultato fine a se stesso, ma lo considerava come un tassello di conoscenza che gli permettesse di trovare l'equilibrio Grazie - e unione con l'ambiente in cui si muoveva. Da questo nasceva la sua profonda conoscenza di questo ambiente e la sua consapevolezza di doverlo difendere dall'intervento devastante dell'uomo. Voglio citare un'altra frase di Maiorca anche per rendere omaggio all'eccellente narratore qual è stato e per farci cogliere ancor meglio la sua unicità. Disse: «Fu un pescatore greco a spiegarmi come il cervello e il cuore dell'uomo fossero molto più sconosciuti degli abissi marini. Per conoscerli davvero bisogna prima conoscere la propria anima e il proprio cuore». Ho voluto ripercorrere questo

di essere un grande esploratore, accumulare conoscenza rispetto a quanto stava facendo e la grande intelligenza e e onestà intellettuale per tradurre ciò che aveva compreso da questa esperienza in un impegno civile. Ha avuto il grande coraggio (badate bene che entrare in politica richiede davvero un grande coraggio)

Grazie

è trasmettere ciò che ha distinto la sua unicità: l'essere stato un campione nello sport, ma anche un campione nella vita, mettendoci di fronte a un specchio che ci ha fatto comprendere in quale direzione deve andare

il testo di quei subemendamenti non ci è stato di fatto consegnato, ma è stato semplicemente letto in Aula. Abbiamo preteso, come è nostro diritto, che quei due emendamenti potessero essere subemendati così abbiamo fatto nel corridoio fuori dalla Commissione, scrivendo i subemendamenti a mano e non avendo neanche il tempo di capire, con la giusta cognizione di causa, cosa stesse avvenendo e quello che stavamo leggendo. Il presidente della Commissione Casini ha affermato che non potevamo entrare nel merito di quegli emendamenti, perché non erano di nostra competenza, essendo emendamenti richiesti dalla Commissione bilancio. A questa affermazione ho obiettato chiedendo

Non è stato possibile effettuare le nostre dichiarazioni di voto, né sugli emendamenti, né sui singoli articoli. Mentre stavamo parlando degli emendamenti e del provvedimento, la Commissione

di parlamentari in generale e di parlamentari membri di una Commissione. In questo momento non sappiamo quale sia la scadenza per la presentazione degli emendamenti in Assemblea e, lo ripeto, non ci è stato consentito di fare una votazione né sui singoli emendamenti, né sul disegno di legge di ratifica nel suo complesso. Quindi chiedo

Presidente, come Presidente della Commissione affari esteri,

peccato per un eccesso di liberalità. Racconto i fatti: nella seduta di questa mattina della Commissione affari esteri, emigrazione - una delle ennesime sedute, perché aspettavamo il parere della Commissione bilancio il relatore ha presentato due emendamenti per soddisfare esclusivamente le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. I colleghi del Movimento 5 Stelle, alle ore 9,15, hanno chiesto la possibilità di subemendare tali emendamenti. Nonostante l'evidente natura ostruzionistica della richiesta, in considerazione la correttezza di rapporto che abbiamo sempre avuto con i colleghi del Movimento 5 Stelle, che peraltro già in apertura di seduta di Commissione avevano posto un problema in ordine alla regolarità delle procedure elettorali del voto degli italiani all'estero, che non è di stretta competenza della nostra Commissione perché - come è noto - come è noto - tale procedura dipende dal Ministero dell'interno per cui ho fatto riferimento alla Commissione affari costituzionali, che sarebbe stata comunque la depositaria di questa eventuale richiesta. per cortesia verso i colleghi, ho investito del problema il sottosegretario Della Vedova e ho detto che se ci fossero stati ulteriori problemi, la depositaria di tali richieste sarebbe stata la senatrice Finocchiaro, quale Presidente della Commissione affari costituzionali. Eppure c'è stato un dibattito su questo aspetto, del tutto improprio, ma tollerato da parte mia e anche della maggioranza, per cortesia verso i collegi del Movimento 5 Stelle. Nonostante l'evidente natura ostruzionistica della richiesta, dunque, alla fine abbiamo ritenuto di concedere tale possibilità. Ho infatti ritenuto importante salvaguardare le prerogative dei parlamentari, contemperandole ovviamente con l'esigenza del buon andamento dei nostri lavori e, in particolare, di quelli dell'Assemblea. Erano le ore 9,20 e ho concesso cinque minuti per la presentazione dei subemendamenti.

i colleghi della Commissione, a riprova dell'intento evidentemente ostruzionistico, hanno chiesto di illustrare gli emendamenti. Ho detto loro che non c'erano i tempi per farlo. Abbiamo dunque regolarmente votato i subemendamenti e gli emendamenti presentati dalla Commissione per adempiere alla prescrizione della Commissione bilancio. Il discorso termina qui. Si trattava di emendamenti auto evidenti, che parlavano l'uno di opportuna rivalutazione del costo dell'opera, l'altro degli oneri non esplicitati nel testo dell'accordo. È chiaro che non c'era alcuna esigenza di illustrazione, visto che dalla semplice lettura tutti i colleghi erano perfettamente in grado di esprimere un voto consapevole. amareggiato per questo comportamento. Capisco che la TAV è un argomento che vi sta a cuore e che vi consente di fare qualsiasi battaglia politica. Le fate linearità emendando gli emendamenti che la Commissione bilancio ci ha chiesto di presentare e che il senatore Sangalli, come relatore, ha presentato. È vostro diritto fare battaglie politiche, però credo che le stesse abbiano un confine nel rispetto delle forme anche tra colleghi e questa mattina francamente non è stata scritta una pagina esaltante.

ne pensa un'altra cosa. Sarà un loro problema. Non lo faccio con i miei e non mi permetto di farlo con i vostri. Ciascun parlamentare, visto che ci attribuiamo uno *status* giuridico molto importante, come è giusto che sia, nel nostro panorama politico italiano,

affari interni (questa è una nota abbastanza simpatica). Possiamo anche sorvolare sul fatto che i membri della Commissione affari esteri sono per la maggior parte eletti nella circoscrizione estero, quindi sono i primi a essere i garanti di determinate prerogative. Possiamo sorvolare sul fatto che i membri della Commissione esteri per la maggiore parte sono anche membri del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, quindi il giudizio di mancata competenza della Commissione affari esteri sollevata da presidente Casini potrebbe anche lasciare

Senatore Lucidi, lei ha avuto tutta la possibilità di prospettare i suoi dubbi e le sue valutazioni. Potrà entrare nel merito nel momento in cui si discuterà in Aula,

Se mai si farà, e questo lo vedremo, perché le situazioni possono cambiare molto rapidamente, soprattutto in Italia. Signor Presidente, le sto chiedendo semplicemente, con estrema cortesia e pacatezza: non ci è stato comunicato il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea; sto sollevando questo problema perché c'è stato chiaramente un problema procedurale in Commissione. Questo è evidente, non possiamo non essere d'accordo su questo. Mentre noi parlavamo, i nostri colleghi votavano. Questo non è un esercizio di grande democrazia.

il fatto che se noi non abbiamo un termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è perché non ci è stato comunicato. La pregiudiziale l'abbiamo presentata ieri, ma i subemendamenti sono stati presentati oggi.

la prego di esercitare tutte le sue prerogative da senatore quando si tratterà di questo argomento in Aula. Adesso abbiamo un altro argomento all'ordine del giorno.

Grazie Presidente, volevo ringraziare lei e il presidente Casini per avere esplicitato in maniera chiara che le obiezioni del collega Lucidi non avevano fondamento e che sono e che sono soltanto un modo di fare ostruzione su un tema che, legittimamente, il Movimento 5 Stelle non vuole sia trattato in Assemblea. Noi però, altrettanto legittimamente, vogliamo dire invece che l'approvazione della

perché crediamo sia uno strumento importante per lo sviluppo di questo Paese e sia anche un modo per dimostrare che l'Italia è capace di tenere fede agli impegni che assume a livello internazionale. Volevo sottoporre all'Assemblea anche l'urgenza di ripristinare, da questo punto di vista, l'ordine del giorno che ci eravamo dati e che era stato

di essere certi che i lavori proseguiranno con speditezza e assoluta trasparenza, senza che vi sia alcuna possibile infiltrazione della criminalità in un'opera così importante,

la trattazione immediata di questo provvedimento. Infatti abbiamo una data molto precisa, il 31 dicembre, entro la quale la ratifica va portata a compimento, anche con una deliberazione dell'altro ramo del Parlamento. Siamo in stagione di

Signor Presidente, io ritengo che il provvedimento che stiamo discutendo, relativo alla responsabilità professionale, sia un argomento altrettanto e più importante rispetto alla questione della TAV. È stato così importante che, concluso il voto degli emendamenti, in Commissione abbiamo votato immediatamente il testo, senza neanche averne una versione scritta, correttamente emendata, per poterlo inserire

Questo era stato sottolineato dalla Commissione igiene e sanità, e questo dimostra che il provvedimento che stiamo discutendo, concernente la responsabilità professionale, è certamente più urgente, anche perché dovrà tornare di nuovo alla Camera. riteniamo che non si debba procedere all'inversione dell'ordine del giorno. *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di conoscere il numero degli otto senatori che hanno richiesto l'inversione dell'ordine del giorno. Dopodiché, prima di proseguire con la votazione per alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

fatto a Parigi il 24 febbraio 2015; *b)* del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti

*relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca ratifica ed esecuzione dell'accordo sottoscritto

ritenuta un collegamento essenziale per la creazione di un efficiente asse di trasporti lungo la direttrice est-ovest del Continente europeo, per consolidare ulteriormente l'interscambio economico fra l'Italia e gli altri Paesi europei, rilanciando il trasporto ferroviario, rispetto a quello stradale, soprattutto per le merci. Secondo i presupposti che stanno alla base del progetto, il Corridoio Mediterraneo, di cui la Torino-Lione è parte essenziale, rappresenta per l'Italia una delle principali reti a supporto del tessuto industriale, perché è in grado di garantire maggiore accessibilità ed una migliore connessione con gli altri corridoi transeuropei che passano per l'Italia. Come Paesi firmatari della Convenzione delle Alpi, l'Italia e la Francia promuovono altresì la sostenibilità ambientale dei trasporti. A tale riguardo è stato stimato che la costruzione della nuova linea essenziale anche in ragione dell'inadeguatezza al trasporto ferroviario moderno della linea storica del Frejus - porterà ad una riduzione annuale di emissioni di gas serra di circa 3 milioni di tonnellate, equivalenti a quelle prodotte da una città di 300.000 abitanti. Si tratta quindi di un contributo importante nell'ambito della strategia europea di riduzione dei gas ad effetto serra come previsto nell'accordo siglato a Parigi nell'ambito della COP21 e recentemente ratificato dal nostro Parlamento. L'Unione europea aveva previsto la creazione di una rete ferroviaria transeuropea già dal luglio 1996, estesa poi nel 2004 ai nuovi Paesi membri. Di questa rete la linea Torino-Lione è un asse prioritario, perché attraversa due delle maggiori aree sviluppate del continente: la zona sudorientale della Francia e la Pianura padana. La linea si inserisce infatti nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti, uno dei dieci corridoi ritenuti prioritari dall'Unione europea. Anche in considerazione del rilievo strategico che le viene riconosciuto, la Torino-Lione ha potuto contare, già in fase di studio, di importanti quote di cofinanziamento europeo. particolare, ha deciso di cofinanziare l'opera sottoscrivendo un accordo di finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per cento dell'ammontare delle spese. Si ricorda che Italia e Francia hanno siglato, nel gennaio 2012, un accordo (esaminato ed approvato anche dalla nostra Assemblea nell'aprile 2014), che ha fissato la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera dell'opera nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 a carico della Francia, al netto del contributo europeo. Con gli accordi al nostro esame si conclude l'*iter* per consentire l'avvio dei lavori definitivi nella sezione transfrontaliera, con il cofinanziamento di cui si è detto. Si ricorda anche che tale sezione costituisce la prima fase di realizzazione dell'opera e si estende per circa 65 chilometri fra le cittadine di Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa/Bussoleno in Italia. Il suo elemento fondamentale è una galleria di 57 chilometri (di cui 45 in territorio francese e 12 in territorio italiano) che consentirà di limitare la pendenza massima dell'attuale linea di montagna esistente fra Torino, Bardonecchia, Modane e Lione e dunque di abbattere del 40 per cento il costo energetico di attraversamento per i treni merci lungo la tratta. Gli *iter* autorizzativi in entrambi i Paesi si sono conclusi nel 2015 ed attualmente è in corso la finalizzazione del cosiddetto progetto di riferimento finale, che recepisce tutte le prescrizioni derivanti dagli atti approvativi nazionali. Vediamo adesso più nel dettaglio i tre accordi al nostro esame. L'Accordo del 24 febbraio 2015 dispone l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria, affidandone la realizzazione al promotore pubblico Tunnel Euroalpin Lyon Turin e rinvia la definizione del costo certificato del progetto ad un protocollo addizionale da definirsi fra i due Paesi. L'Accordo riafferma l'impegno della parti a lottare contro i tentativi di infiltrazione mafiosa (articolo 2), disciplina altresì aspetti relativi all'organizzazione della committenza dei lavori connessi (articolo 4), alle modalità di funzionamento del promotore pubblico (articolo 5). Il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016, composto di una premessa e di quattro articoli, ha per oggetto la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori. L'articolo 2, in particolare, quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e definisce la relativa ripartizione fra le parti. Il paragrafo 2.1 prevede nello specifico che le parti assumano un costo certificato. L'attualizzazione è soggetta a verifica annuale fino al completamento dei lavori, sulla base di un apposito indice di riferimento. Il Regolamento dei contratti, definito dall'apposita Commissione intergovernativa, ha per oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti, sia quelli conclusi dal promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori o subaffidatari. Il Titolo III disciplina i motivi per escludere le imprese dalla partecipazione, diretta o indiretta, alle procedure per la realizzazione dell'opera. Ad un'apposita commissione mista viene delegato il compito di assicurare il funzionamento dei meccanismi di prevenzione del rischio di infiltrazioni o condizionamenti criminali, tra cui una «Lista bianca» degli operatori economici nei cui confronti non siano emerse situazione ostative. Di rilievo è altresì l'articolo 12, che disciplina il tracciamento e il monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ai contratti per la realizzazione dei lavori. Attraverso il Regolamento dei contratti si realizza dunque l'integrazione della normativa italiana nel *corpus* giuridico francese in materia di contratti pubblici. Con la ratifica dell'Accordo in esame da parte del Parlamento francese, tale Regolamento, in quando atto di diritto internazionale, ha un valore giuridico prevalente rispetto alla legge ordinaria. Ci sono quindi precise garanzie circa l'esclusione di possibili infiltrazioni mafiose nella realizzazione dell'opera. Peraltro il Regolamento dei contratti, che non costituisce un atto autonomo e distinto dall'Accordo del 2015

appare inoltre del tutto conforme a quanto statuito dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto in materia di trattati. Ci sono del resto dei precedenti esempi di trattati internazionali per i quali il Governo francese ha delegato ad apposita commissione bilaterale il compito di redigere norme di natura legislativa o regolamentare immediatamente valida per l'ordinamento interno. È già accaduto per la definizione delle norme in materia di concorrenza e sicurezza ferroviaria per il Tunnel della Manica nel 1986 e per il Tunnel del Monte Bianco nel 2006. Contrariamente a quanto sostengono alcuni critici del progetto quindi, l'applicabilità della normativa antimafia italiana anche nell'ordinamento francese non è assolutamente controversa. Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, circa l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le modalità realizzative dell'opera e l'entrata in vigore del testo. In relazione agli aspetti tecnico-finanziari, la relazione evidenzia come per la realizzazione dell'opera si provvederà, a legislazione vigente, per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le Parti nei soli limiti di finanziamento che il Governo renderà effettivamente disponibili, in coerenza con il cronoprogramma dei lavori. con il cronoprogramma dei lavori. L'articolo 2 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CIPE deliberi in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse già disponibili a legislazione vigente, che ammontano a 2.564,7 milioni di euro. Il medesimo articolo quantifica in poco più di 25.000 euro il totale degli oneri derivanti dal Regolamento degli oneri derivanti dal Regolamento dei contratti, ascrivibili a spese di missione per i membri della struttura binazionale paritetica, nonché per l'effettuazione di visite ispettive nei cantieri di lavoro. In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame. *(Applausi Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale. Ha chiesto di intervenire il senatore Lucidi per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dare una breve risposta al senatore Russo; la Commissione bilancio è stata forzata a discutere il parere su questo emendamento, come al solito, per una manovra del Governo che impone la sua azione sul nostro Parlamento e questo dovrebbe essere un punto di estrema riflessione per noi. Non ci dimentichiamo che però la Commissione bilancio in queste ore sta trattando i due famosi provvedimenti sul terremoto. Non credo che ci sia una lotta di urgenza su questo tema. Non è questo sicuramente che gli italiani stanno aspettando. Detto questo, entriamo nel merito. Stiamo discutendo il disegno di legge n. 2551, che reca l'autorizzazione alla ratifica alla ratifica di due atti: il primo è l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015.

Esaminiamo nel dettaglio il provvedimento che stiamo andando a ratificare. L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica di entrambi gli atti che ho citato poco fa, ma così facendo, come è già accaduto molte volte purtroppo, i membri del Senato non potranno esprimere il proprio voto in maniera difforme tra il primo e il secondo atto.

prevedente l'approvazione del disegno di legge con votazione articolo per articolo, prima in Commissione e poi in Assemblea - non permetterà ai Senatori di esprimersi, a mero titolo d'esempio, favorevolmente sul Trattato il disegno di legge in titolo reca proposta di ratifica dei suddetti trattati bilaterali in attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con i relativi Allegati. L'Accordo citato, a sua volta, rappresenta espressamente il «protocollo addizionale» dell'Accordo quadro del 2001.

la Repubblica francese, in particolare la Commissione mobilità 21, istituita presso il Ministero dell'ambiente, ha escluso, nella sua relazione finale, di procedere ai raccordi alle linee esistenti, poiché linee esistenti, poiché «date le incertezze sul calendario del tunnel di base, la Commissione non è stata in grado di garantire che il rischio di saturazione della linea e del conflitto sulla linea che giustificherebbero la realizzazione del progetto avverrebbe prima del 2035-2040».

di non procedere a successivi accordi: «date le incertezze sul calendario del tunnel di base, la Commissione non è stata in grado di garantire che il rischio di saturazione della linea e del conflitto sulla linea che giustificherebbero la realizzazione del progetto avverrebbe prima del 2035-2040». Ciò significa che questa Commissione sta classificando il progetto di accesso al collegamento binazionale Torino-Lione come seconda priorità indipendentemente dallo scenario finanziario considerato. Ciò rilevato, occorre ricordare che ogni condizione che infici il primo atto, di cui al comma *a)*, determina la nullità del secondo; questa condizione - la ratifica di un accordo ineseguibile - costituirebbe già di per sé una palese dell'articolo 97 della Costituzione che impone il buon andamento della pubblica amministrazione. Ma c'è anche altro. Italia e Francia il 24 febbraio 2015 hanno sottoscritto l'Accordo di cui alla lettera del primo capoverso del presente documento, «per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione». Detto Accordo prevede un Protocollo addizionale, composto da quattro articoli, avente medesimo oggetto e da concludersi «a mezzo scambio di lettere». Concordiamo su questo punto, onorevoli colleghi? L'accordo prevede un Protocollo addizionale composto da quattro articoli, avente medesimo oggetto e da concludersi «a mezzo scambio di lettere», ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo medesimo,

dell'Accordo del 24 febbraio 2015. Quindi il Protocollo risulta siglato congiuntamente, in modo similare all'Accordo. Non so se è chiaro il concetto. Ancora più nel dettaglio, il citato articolo 3 dell'Accordo definisce il «costo certificato del progetto a valuta gennaio 2012». Quindi siamo già quattro anni oltre la valutazione fatta e citata all'articolo 3 dell'Accordo. Detto costo è «validato», come accennato al capoverso precedente, tramite il Protocollo addizionale che si intende ratificare contemporaneamente all'Accordo;

istituzionale o burocratico. Lo scambio di lettere, che avrebbe dovuto concludere l'Accordo, in realtà non si è verificato. E questo è un altro punto - secondo me importante - che osta

Veniamo ora all'articolo successivo, l'articolo 5, dell'Accordo del 24 febbraio 2015, che emenda l'Accordo siglato nel 2012, che rappresenta la fonte normativa atti pattizi che si intende ratificare tramite il disegno di legge in titolo. In particolare, l'articolo 7.5 dell'atto è modificato prevedendo che «la commissione dei contratti pronuncia il proprio parere entro i tempi minimi possibili e comunque non oltre i 90 giorni». In precedenza era citato solo il termine di novanta giorni.

le nostre motivazioni ostative all'approvazione del disegno di legge in esame. C'è un fatto importante, che ho citato prima: in realtà c'è un altro Stato. Molto spesso noi, senatore Russo, facciamo riferimento ad ad altri Paesi come modelli, ma purtroppo lo facciamo, o meglio lo fate soltanto quando vi conviene o vi fa comodo. Quando il riferirsi a modelli esteri, e quindi a modelli esterni rispetto al nostro ordinamento, potrebbe essere invece una scelta di buon senso e logica, non lo fate. Comunque sia, per tutti i motivi che ho parzialmente espresso nel corso di questa mattinata, e non soltanto in questo intervento, ma anche in quello precedente, e per quelli contenuti nella nostra proposta di questione pregiudiziale, chiedo che l'Assemblea deliberi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non

indonesiano che, nel secondo ordine di tribune, sta seguendo i nostri lavori. Benvenuti in Italia, benvenuti al Senato della Repubblica.

Signor Presidente, noi voteremo a favore della questione pregiudiziale testé illustrata dal senatore Lucidi

alle regole applicabili al fine di contrastare e prevenire le infiltrazioni criminali mafiose. italo-francese del 2012 per la realizzazione della linea Torino-Lione, che è collegata all'atto che stiamo esaminando, ha un protocollo particolare per quanto riguarda la realizzazione e la futura gestione della sezione

al massimo prevede l'uniformazione degli *standard* - e questa è la seconda balla che viene continuamente raccontata in questa Assemblea. In terzo che il traffico merci ha bisogno di una nuova linea ferroviaria, e questo è stato già ampiamente dimostrato. Persino il Politecnico di Torino, a cui è stato chiesto di elaborare una valutazione, ha detto

che è pur vero che ci sarebbe una leggera diminuzione dei costi di gestione per la minore pendenza e la minore quota da raggiungere, ma linea ferroviaria andrebbe refrigerata. Questa è la famosa "genialata" di cui non parlate mai. La temperatura nel cuore del *tunnel* sarebbe così elevata da richiedere costantemente l'uso di condizionatori,

meno? Queste argomentazioni sono le stesse che hanno condotto due grandi compagnie aeree, negli anni Sessanta, a pensare di costruire un nuovo aereo, il Concorde,

A un certo punto la necessità di trasportare documenti da un capo all'altro dell'emisfero è venuta meno, perché era più semplice inviarli via *fax* e, quindi, nessuno aveva più voglia di spendere tutti quei soldi... *(Brusio)*.

Per di più nessuno fa la seguente, semplice, osservazione: un treno ad alta velocità e a pieno carico spende il 91 per cento della propria energia per spostare se stesso, e cioè il treno, e solo il 9 per cento dell'energia per spostare i passeggeri. Questo non è un utilizzo intelligente dell'energia, perché la maggior parte di essa viene impiegata per spostare il mezzo stesso. Oltretutto, le previsioni di traffico passeggeri su quella linea ci

a una crisi del commercio mondiale e al fallimento della sesta più grande compagnia di trasporto marittimo, che senso ha pensare a un'opera di trasporto merci totalmente svincolata dal contesto mondiale? Ovviamente non ha senso. Dobbiamo dire anche un'altra cosa: pensiamo al trasporto merci. Vi ricordate? Non esistono carri ferroviari per il trasporto merci ad alta velocità, né sono allo studio: vanno a 90 o, al massimo, a 120 chilometri orari. Nel momento in cui inserite tracce orarie all'interno di un percorso alternando mezzi che dovrebbero andare a 300 con altri che dovrebbero andare a 90, spiegatemi dove è l'economicità dell'operazione. Ovviamente non c'è.

a circa 37 chilometri orari, improvvisamente dovrebbe recuperare il tempo perso balzando su un treno e venendo trasportato ad alta velocità,

che va in Europa ad alzare la voce dicendo che forse porrà il veto dopo aver votato per 148 volte su 148 a favore di ogni provvedimento della Commissione europea, domanda. Visto che sta andando a piangere miseria per poche centinaia di milioni, perché ha intenzione di impegnare miliardi di risorse in questa opera che non si ripagherà mai? La società Eurotunnel insegna: non è mai stata in pareggio e non ha mai prodotto un centesimo di utile; è continuamente ricapitalizzata da Francia e Gran Bretagna. Eppure, è in completa saturazione. Questa opera non funziona da alcun punto di vista. Prima di trovarci con l'elefante bianco, sarebbe meglio fermarsi e non impegnare risorse in questo.

se i soldi che spendiamo hanno un beneficio per la collettività. Come abbiamo detto tante volte, la linea storica non è satura; anzi,

merci. Noi abbiamo speso 400 milioni di euro per adeguare un *tunnel* che già esisteva. Ora vogliamo spendere una cifra molto elevata di soldi dei contribuenti

minuti. Spendiamo 6 miliardi di euro per risparmiare venti minuti nella vita di un pomodoro. Non è una cosa da poco. Anzi, mi sembra molto importante per fare bene le pizze francesi.

Frejus. Se queste sono le situazioni sulle quali ci troviamo a ragionare, ci volete spiegare a che serve fare il buco? È questo il vero dramma. Poi ci sono anche degli aspetti tecnici: leggiamo nella relazione che il progetto definitivo è stato approvato nel febbraio 2015.

perché spendiamo tutti quei soldi? Ecco, adesso mi viene in mente: forse il Governo si è innamorato di quel signore che, con una borsetta, diceva: «L'economia gira con te». Spendi i soldi, così facciamo il bene del Paese.

resistenza - come è stata spesso chiamata - dei cittadini della valle, che semplicemente si sono visti imporre senza alcun dialogo un'opera inutile,

perché i vostri *partner* internazionali non erano molto convinti; perché quest'opera costa oggettivamente troppo; perché il problema in Italia è fondamentalmente la corruzione che appesta le amministrazioni, i progetti, i vostri partiti, questo Governo e quello precedente ancora. Ve la siete presa con un popolo. Una volta un giornalista mi ha chiesto quanto fosse lecito che i valsusini si ribellassero a un'opera. Ma la domanda vera sarebbe stata: quanto è lecito che uno Stato con arroganza e svilendo qualsiasi rapporto democratico metta le mani su un territorio

questo incredibile e inaudito progetto di violenza nei confronti di un popolo al quale non avete mai avuto neanche il coraggio di parlare. Avete fatto fare gli osservatori a dei signori che sono stati pagati per non fare nulla.

Non c'è mai un dialogo. Non c'è mai la possibilità di confrontarsi in quest'Aula, per capire perché buttare via decine di miliardi, quando il Paese va a fondo, in un'opera che non siete stai mai capaci di fare. Avete iniziato con un *tunnel* geognostico e poi avete cambiato progetti. Il popolo valsusino vi ha interpellato in tutti i modi possibili e non solo, ed è riuscito a uscire dalla Valle, a

non puoi opporti e magari ti fa un *tunnel* in casa o ti pianta una trivella in salotto. Può essere una battuta? No, e non lo è perché quando andammo da Caselli a mostrargli le criticità del primo accordo, i

- Sala si lamenta e chiede l'intervento dell'esercito per garantire la sicurezza. Peccato che i militari e gli alpini, che spesso vediamo agli angoli delle piazze, non possano garantire l'ordine pubblico, perché non sono autorizzati, o possono farlo ma molto limitatamente. Ora, vorrei far notare che

una vera responsabilità che pesa su di voi. E io vi assicuro che, quando ci ritroveremo qua, o fuori di qua, e questa opera non sarà stata realizzata, dovrete ammettere che avete fatto veramente pena, che siete stati vergognosamente servi esclusivi di una classe corrotta, di amministratori, di progetti, di multinazionali e di un potere europeo che ormai vi guida come burattini.

Infatti, oggi la rappresentazione chiara del nostro Paese è che siamo estremamente competitivi per quanto riguarda l'alta velocità, in ambito internazionale ed europeo,

italiane, con grande successo, e poi dire che a casa nostra non vanno bene. A casa nostra bisogna fare chiarezza su determinate determinate filosofie e determinate visioni per quanto riguarda la ferrovia. Credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che, se vogliamo togliere dalle

candidamente che la privatizzazione delle ferrovie era solo un sistema per far cassa (lo ha detto lui). Dunque: mettetevi d'accordo! Dal nostro punto di vista, sposando la filosofia per cui chi semina strade raccoglie traffico, dobbiamo guardare i Paesi che sanno fare i progetti seriamente, bisogna realizzare le ferrovie e farlo con certe condizioni ed è del tutto evidente che la privatizzazione e tutte le azioni che vanno sul grande sistema di trasporto ferroviario sono un'occasione di rilancio e di sviluppo per il nostro Paese. Ora, se guardo alla programmazione che c'è in questo momento al Ministero delle infrastrutture e dei

esserci tutto un sistema integrato che favorisca le condizioni sia per il trasporto merci che per il trasposto ad alta velocità dei passeggeri che deve essere conseguentemente agganciato. Noi più volte abbiamo dato stimoli a questo Governo affinché le adduttrici ai grandi trafori alpini, nel nostro Paese e al di fuori, siano compiute nel più breve tempo possibile. Infatti, se vogliamo ricevere quei 700 treni al giorno che potrebbero vomitarci da AlpTransit dobbiamo essere preparati, collega Della Vedova: dobbiamo fare le adduttrici, che sono che sono le ferrovie che salgono sulla sponda orientale del lago Maggiore, dobbiamo potenziare la linea Milano-Chiasso e dobbiamo fare le adduttrici anche per la TAV. Questo per cercare di essere un minimo competitivi con i 73 chilometri di banchina che ci sono al porto di Rotterdam, ovvero con un sistema di trasporto

noi. Mi rivolgo ancora ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Sanno benissimo anche loro che la Confederazione Elvetica ha messo sul piatto importanti finanziamenti affinché il nostro Paese si decida a fare, con Hupac o con altri sistemi, un un sistema integrato in cui le merci possono scendere verso sud ed essere trasportate sulle autostrade del mare. Noi dobbiamo pertanto assolutamente perseguire questa

Ministeri: mettetevi d'accordo su di che morte volete morire. È un dato di fatto che, dal punto di vista strategico, il nostro Paese deve assolutamente

500 metri. Sono due cose completamente diverse. Se facciamo i trafori di base dei grandi valichi alpini è perché vogliamo delle ferrovie

forse c'è ancora un po' di confusione nella testa di qualcuno. Queste sono le condizioni sulle quali dobbiamo lavorare e le prerogative ci sono. Ribadisco, come dirò in dichiarazione di voto, che noi siamo favorevoli: l'unica preoccupazione è che il Governo anche su questa partita sia in stato confusionale. nostra intendiamo continuare in questa direzione, perché è un progetto che avete ereditato ed è un progetto serio con il quale il nostro Paese si è presentato in ambito europeo e, se non sbaglio, entro il 31 dicembre dobbiamo riscuotere il 40 per cento dei finanziamenti europei, perché altrimenti ci giochiamo anche questi.

Devo dire però brevemente che il caso del Gottardo è assolutamente un'altra cosa rispetto alla linea Torino-Lione: ci sono totali diversità sia logistiche che trasportistiche per quanto riguarda le merci e comunque nessuna componente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha mai fatto neanche un *tweet* di elogio di questa grande opera svizzera (ricordo: svizzera, perché qualcuno ha ancora dei dubbi)

Tornando a noi, devo ammettere che la tentazione di insultarvi per venti minuti era tanta, ma avrebbe avvalorato l'ipotesi che il Movimento 5 Stelle riesca solo a insultare e non a proporre e a entrare nel merito delle cose,

vi siano ancora troppi corpi caldi in giro sul nostro territorio, mentre qui si fanno azioni politiche per mandare avanti una grande opera, probabilmente per paura che il prossimo mandato governativo tolga ad alcuni amici le prebende che sono state promesse. Questo è inutile dirlo, perché voi lo sapete benissimo. Tutti i provvedimenti importanti sono fermi, si basano solo sulle parole del *Premier* e non sono mai stati seguiti da atti, come sempre: rimangono mere parole che sanno di presa in giro. In questa infinita storia,

un'idea, sbagliata, che nulla ha a che vedere con la democrazia. Detto questo e confermato, quindi, il "disonorevoli senatori", questa mossa è altamente inopportuna. Mio malgrado e con il disagio di dover sedere nella stessa stanza in cui voi vi trovate, passo in rassegna alcuni punti critici, per buona parte anche incostituzionali o, se vogliamo, truffaldini di questi trattati. Ovviamente, voi li ratificherete senza neanche battere un ciglio. Sono due: Sono due: l'Accordo e il Protocollo addizionale che, a detta dell'Accordo, dovevano essere approvati separatamente, mentre voi li state approvando insieme. Primo punto. L'Unione europea non ha definito la piena partecipazione al progetto, né ha quantificato la percentuale di finanziamento dello stesso, quindi vi è indeterminatezza dei costi. Come specificato nell'articolo 1 dell'Accordo del 2012, l'Accordo stesso non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo del 2001 precedentemente citato e, in particolare, non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo addizionale opzionale separato (appunto: separato), tenendo conto, in particolare, della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto (articolo 1, La deliberazione CIPE del 20 febbraio 2015, n. 19, ribadisce, alla quartultima riga delle premesse, che l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese resta, infatti, subordinato

l'energie assegna un contributo di circa 814 milioni di euro, a fronte di spese programmate per circa 1,9 miliardi di da realizzarsi entro il 31 dicembre 2019. Le attività alle quali l'Unione europea ha assegnato l'attuale contributo riguardano sia i lavori preliminari, ma difficilmente i lavori definitivi potranno essere completati, tenuto conto che nel Grant agreement, all'articolo 1, comma 3, si specifica che gli studi in corso e le indagini geologiche saranno completati aprendo la strada per i lavori preparatori e l'inizio delle principali opere civili, che proseguiranno oltre il 2019 fino al loro completamento. Pertanto, l'azione è una fase intermedia di un investimento complessivo di infrastrutture in questa regione. Appare quindi evidente che il programma sul quale l'Unione europea ha assegnato il contributo consiste in una spesa drasticamente inferiore, pari a circa 1,9 miliardi, rispetto a quella necessaria per la realizzazione del progetto della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria, il cui costo, ai sensi del Protocollo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è stimato intorno agli 8,3 miliardi Se ne deduce quindi chiaramente che il contributo europeo assegnato con il *Grant agreement* non definisce la partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto, in quanto non riguarda la realizzazione complessiva del progetto stesso. Infatti, eventuali ed ulteriori future partecipazioni dell'Unione europea potranno verificarsi soltanto a seguito dei seguenti passaggi: assegnazioni di fondi nel bilancio dell'Unione europea; successiva emissione di bandi dedicati al finanziamento di grandi infrastrutture di trasporto transfrontaliero; presentazione da parte dei Governi italiano e francese di specifiche domande di finanziamento; eventuale accettazione di tali domande e assegnazione dei relativi finanziamenti. Il tutto da spalmare sulle prossime legislature dell'Europarlamento, per avere un po' più di fondi che ovviamente non ci sono. Nessuno dei passaggi sopraelencati è ad oggi garantito o assicurabile, in quanto nessuna istituzione europea ha la possibilità di vincolare per il futuro i bilanci dell'Unione. dell'Unione. Ciò detto, ne consegue che a tutt'oggi non sussistono le condizioni esplicitamente richieste dall'Accordo del 2012 e dalla delibera CIPE 19/2015, ai sensi dei quali è richiesta partecipazione definitiva dell'UE a questo progetto. Quindi, come affermato, è chiaro che attualmente una ratifica dell'Accordo del 2015 e del Protocollo aggiuntivo del 2016 che è in esso contenuto si pongono in diretto contrasto con l'Accordo del 2012 e con la delibera CIPE 19/2015. Eppure ve ne fregate, ma questo noi lo sapevamo già: dopo il mostro giuridico della "schiforma" Boschi, per voi queste sono bazzecole, quisquilie, pinzillacchere. Passando

nella parte che disciplina la commissione dei contratti, composta da dodici membri nominati per metà da ciascuna parte con scambi di lettere tra le medesime parti potete nominare la commissione mandandovi delle lettere? Ma stiamo veramente scherzando? - in tal modo permettendo che gli eventuali emendamenti proposti sfuggano alla valutazione e alla successiva ratifica parlamentare. La riforma costituzionale abolisce in parte il bicameralismo, che era perfetto, ma questo accordo abolisce direttamente tutto il Parlamento: si faranno emendamenti con scambi di lettere. Tutto questo è veramente ridicolo, alla faccia della Repubblica parlamentare e della democrazia! Le parti modificabili attraverso scambi di lettere intervengono, tra l'altro, su ambiti rilevanti, quali i criteri preposti alla selezione delle candidature e delle offerte, la validità dell'eliminazione delle candidature e delle offerte, nonché i mezzi materiali e finanziari a disposizione della commissione dei contratti, necessari a permetterne il corretto funzionamento, ovvero, come si suol dire, dove c'è la ciccia, dove ci sono i soldi e dove si può fare un favore a un amico piuttosto che a un altro, dove ci si spartisce la torta. Inutile negarlo: è successo per il terzo valico, dove sono stati pizzicati con le mani nella marmellata, e succederà anche qui prima o poi (finora è andata bene per qualcuno); ma, come vedremo più avanti, questa volta gli fornite precisi strumenti per nascondersi e per non essere neanche individuati mentre vanno all'incasso. Andando oltre, all'articolo 6, del tutto inopportunamente, si ribadisce il trasferimento al promotore pubblico del ruolo di gestore di infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane e del tratto relativo alle interconnessioni di Avigliana e Bussoleno con la nuova linea. In pratica, state dando a una società di diritto francese una tratto di una linea italiana, attualmente in gestione a RFI: oltre alla sovranità della nazione, anche le infrastrutture state dando agli esteri. Per quali motivazioni? Perché una linea che fino al confine è ora sotto il controllo di RFI deve invece passare sotto quello pubblico? Per quale motivo? Quali sono le regole che dovranno essere rispettate? Chi garantirà poi la sicurezza di quella linea? Dopo voler fare ammalare i cittadini valsusini con un'opera devastante, che va comunque a toccare delle importanti falde della montagna, volete anche devastarli e annientarli con incidenti ferroviari? Passiamo al Protocollo, al Protocollo, la seconda parte dell'Accordo in agenda oggi. All'articolo 2, comma 2, si prevede un'attualizzazione delle spese di realizzazione a fine lavori. Tale attualizzazione ha lo scopo di effettuare l'adeguamento finale degli scostamenti rilevati, da verificare annualmente mediante un indice di riferimento definito dal protocollo stesso (allegato, punto 3), che consiste in un indicatore di variazione dei prezzi riferiti alle differenti componenti del costo dell'opera. Tale indice, denominato INLTL, deve essere determinato analiticamente secondo le modalità di calcolo stabilite nel Protocollo stesso (allegato, punto 3.1). Per quanto concerne le modalità di aggiornamento dei costi sul lato francese, il Protocollo precisa dettagliatamente, per ciascuna categoria di spesa, il relativo indice di riferimento assunto, precisandone tipologia, fonte e quant'altro. Ma, si sa, in Francia sono precisi, noi invece siamo un po' caciaroni. Infatti, per i costi del lato italiano il protocollo non contiene alcun riferimento certo, limitandosi a generiche e ambigue indicazioni quali: «Per la parte italiana, vengono utilizzati indici analoghi che comprendono le stesse componenti sulla base degli indici italiani» «Per l'ISTAT, gli indicatori rilevati corrispondono il più possibile agli indicatori INSEE e in caso di indisponibilità, agli indicatori equivalenti con un livello di precisione appena inferiore». Ma di cosa stiamo parlando? È evidente che nell'attuale formulazione del Protocollo i criteri di attualizzazione dei costi dei lavori sul lato italiano risultano sostanzialmente indefiniti e mi stupisce che la Commissione bilancio abbia potuto avallare questo. Questa imprecisione, questa precisa e cosciente indeterminatezza creata ad arte per lucrare sull'opera determina un notevole pregiudizio alla corretta applicazione della ripartizione dei costi a fine lavori

potessero essere poi chiamati a risarcire in solido tutte le spese *extra* dovute a questa indeterminatezza che oggi hanno avallato! E non è escluso che, nel caso in cui il Movimento 5 Stelle vada al Governo, questo non avvenga. Quindi, non datevi alla macchia, ma rimanete in zona, perché vi verremo a cercare.

Il predetto articolo 18, però, prevede che il costo stimato del progetto definitivo venga certificato da un terzo esterno. Nel Protocollo non vi è invece alcun riferimento alla certificazione dei costi a opera di un terzo esterno. In ogni caso, la certificazione prodotta dalla Tractebel Engineering è tutt'altro che definitiva e assodata, tenuto conto che a pagina 15 del documento di certificazione si dichiara testualmente: «D'altronde, se la soluzione alternativa sarà prescelta, gli studi futuri consentiranno di chiarire il progetto delle nuove opere e delle opere modificate e di perfezionare la stima attuale del costo e delle tempistiche di costruzione», generando così un'ulteriore indeterminatezza sui costi stessi dell'opera ripartizione tra Italia, Francia e Unione europea e, in ultima analisi, sul bilancio dello Stato per i prossimi anni. Anzi, per le prossime generazioni. A conferma dell'approssimativa stima dei costi dell'opera, appare opportuno segnalare anche quanto affermato nella nota tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in risposta alle osservazioni del relatore, in cui si chiarisce che «Eventuali incrementi del costo certificato previsti dall'articolo 2 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 24 febbraio 2015, saranno oggetto di appositi provvedimenti normativi». provvedimenti normativi». Ma voi avete comunque calcolato le coperture. Fare carte false o chiudere gli occhi pur di approvare questa ratifica infame non vi fa veramente onore. Qui si favorisce chi gonfia i costi, si favorisce chi lucra sulle grandi opere, si favoriscono gli amici degli amici, omettendo, nascondendo e facendoci assistere all'ennesima melina in Aula: di male in peggio. Inoltre, sempre all'articolo 2, viene stabilito che: «Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5

ho detto, mi auguro in futuro possa essere pagato con i vostri soldi, non con quelli dei cittadini, che purtroppo ne hanno sempre meno.

nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera», conferendo «alla commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un regolamento dei contratti» in materia di antimafia. Ed ecco che, con modalità del tutto singolari quanto improprie (per usare un eufemismo), sia l'Accordo che il Protocollo producono effetti giuridici internazionali, ossia l'elaborazione di un regolamento dei contratti prima ancora che i predetti atti siano ratificati e vigenti nell'ordinamento italiano, con ciò facendo sì che il Parlamento esamini un atto, il regolamento, prima ancora che le fonti del medesimo atto vengano ratificate. Vi state rendendo conto che siamo di fronte ad atti consequenziali che entrano in vigore gli uni sulla base degli altri, anche se

sa, per i senatori di questa legislatura va bene tutto: l'importante è servire il capo, la legge non conta più, conta solo assicurarsi una calda sedia per il futuro. Ma il vento cambierà, non vi preoccupate. State molto attenti. Infine, con riferimento al regolamento, va osservato che esso ha ad oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa e di superare il problema dell'impossibilità di effettuare i controlli antimafia riferiti agli appalti, rilevata da più parti, ad esempio anche dal presidente Ma è chiaro come la procedura di ratifica sia inidonea a rendere operative, mediante lo strumento del regolamento, in luogo della modifica dei trattati, le norme italiane antimafia relative sia ai contratti pubblici conclusi dal promotore

di chi vuole arricchirsi, votate quest'opera senza cognizione di causa, ecco che i nostri cugini d'oltralpe risultano ancora una volta un pochino più intelligenti, perché vanno a specificare molto bene tutti i passaggi. Il 10 giugno 2016, il primo presidente della Corte dei conti francese ha indirizzato una comunicazione al primo ministro Manuel Valls in merito alla gestione dell'Agence de financement des Nel rapporto, il presidente Migaud si è mostrato severo nei confronti della gestione, della *governance* e sulla situazione contabile dell'Agenzia, incaricata di allocare i finanziamenti pubblici necessari per la realizzazione delle grandi infrastrutture nazionali, inclusa la quota francese della Torino-Lione. In particolare, la Corte ha evidenziato che la gestione dell'AFITF sarà ancora meno sostenibile sotto il profilo finanziario in caso di realizzazione di nuovi grandi progetti quali la linea Torino-Lione, tenuto conto che il finanziamento del progetto, al di là dell'ipotesi di cofinanziamento europeo, è, in termini di *budget*, ampiamente fuori dalla portata dell'Agenzia, sia con riferimento al 2019 che più in là nel tempo. Badate che l'intervento della magistratura contabile transalpina si inserisce in un percorso di progressivo e radicale ripensamento delle politiche del trasporto ferroviario in Francia, che ha raggiunto il proprio culmine in tempi recenti: il 22 aprile 2013 il Governo francese ha infatti pubblicato le raccomandazioni della missione Bianco, incaricata dall'Esecutivo di stilare linee guida per il futuro dei trasporti su ferro, dalle quali si evince il disinvestimento da nuove linee ad alta velocità. Chissà come mai.

anche se ormai non ci credo neanche più - che il Senato blocchi questo abominio legislativo internazionale. L'Italia ha bisogno di ben altre cose, rispetto a questa linea, che non ha alcun senso di essere realizzata, perché

Come ho detto, illustrando la mia relazione, oggi ci occupiamo della ratifica di un accordo tra Italia e Francia attinente alla costruzione della

Tutto ciò che è stato detto è ovviamente frutto di opinioni diverse. Questa Assemblea e tutto il Parlamento hanno avuto modo di confrontarsi sull'opera, sulla sua utilità e sulle sue caratteristiche

nell'accordo in esame sono state ampiamente adottate in altri trattati internazionali. Certamente, la Francia le ha applicate, acconsentendo anche all'assunzione della legislazione del Paese con cui realizza l'accordo come prevalente rispetto alla propria legislazione nazionale. Dico questo perché la normativa antimafia entrerà nel regolamento dell'accordo, diventandone parte sovraordinata rispetto alla legislazione francese e ciò è avvenuto con modalità identiche

di quest'opera è nota ed è quella di collegare il traffico delle merci ad una direttrice europea ad altissima intensità di produzione la linea attuale, adeguata per entrare in questo ambito. Si collegano alcune delle aree più industrializzate d'Europa e i margini di crescita economica di questa operazione,

l'Accordo prevede una quota complessiva di intervento pari a circa 8,3 miliardi di euro; la quota di competenza dell'Italia è di circa 2,9 miliardi di euro, 2,9 miliardi di euro, la quota di competenza dell'Unione europea è di circa 3,3 miliardi di euro, quella di competenza della Francia è di circa 2,87 miliardi di euro. L'elemento che ha interessato maggiormente il lavoro della Commissione è la compatibilità tra le due legislazioni e l'assunzione nella legislazione corrente francese di tutte le nostre norme antimafia. da verifiche che abbiamo fatto approfonditamente, corrisponde esattamente alla realtà. Questa opera

opererà sulla base di un regolamento che diventa norma sovranazionale. Crediamo che questa ratifica debba essere fatta nei tempi dati, perché questo consentirebbe di essere in regola

La Presidenza dichiara inammissibili l'emendamento 1.3, in quanto privo di reale portata modificativa, nonché gli emendamenti da 1.103 da 1.103 a 1.110, in quanto volti a condizionare la ratifica di un accordo già sottoscritto. In relazione alle modifiche approvate in sede referente per soddisfare le condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio,

gli emendamenti presentati rappresentano il minimo sindacale, perché su un disegno di legge di ratifica si può fare poco. Essi mirano a darvi l'ultima possibilità per evitare questo scempio giuridico. La questione, come ho detto, è che i protocolli aggiuntivi devono essere approvati in maniera separata dall'accordo vero e proprio, e in maniera conseguente e successiva, e che i costi di questa

Per quanto riguarda la questione della legislazione antimafia, mi sembra che, come già detto, un regolamento *inter partes* non possa assolutamente essere considerato un testo di legge vigente in un Paese straniero.

Presidente, intervengo solo per ribadire il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento in esame, sottolineando che in questa fase sarebbe stato assolutamente necessario che il Governo facesse sentire, anche in ambito europeo,

che era stato già stato scritto il 29 gennaio 2001 e ratificato con la legge n. 228 del settembre 2002. Oggi l'Accordo si concentra sostanzialmente sul regolamento, sui contratti e la normativa antimafia, la certificazione dei costi dell'opera e l'aggiornamento del piano finanziario. L'Italia si era impegnata a ratificare l'Accordo entro il gennaio 2017, data che l'Unione europea ha definito tassativa per sbloccare i finanziamenti comunitari a favore della nuova linea ferroviaria.

per presunti episodi di corruzione nei contratti di subappalto ha mostrato ancora una volta quello che noi di Sinistra Italiana e SEL abbiamo sempre denunciato: c'è un verminaio strettamente collegato al sistema delle grandi opere,

l'inaugurazione e il termine dei lavori con il trucco squallido di anticipare la fine della tratta. Quindi inaugureremo il termine della Salerno-Reggio Calabria, ma non è vero: è un clamoroso falso. In passato, di fronte alle responsabilità del Governo nel sistema tentacolare della corruzione in tutta Italia, dall'alta velocità alle autostrade (con i soliti noti coinvolti, quali il *dominus* Incalza, il superdirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o Stefano Perotti, direttore dei lavori della metro C di Roma), avevamo chiesto un taglio netto con le pratiche in uso per archiviare definitivamente la legge obiettivo, madre delle ventennali - e allo stesso tempo quotidianamente rinnovate - pratiche corruttive. Sulla stessa TAV sono intervenuto in più occasioni: un'opera, come molte altre, portata avanti in spregio alla volontà dei cittadini dei territori della Val di Susa, addirittura militarizzata

pericolosa, oltre che costosa e inutile per il futuro del Paese, di impatto devastante. Mi riferisco, solo a titolo di esempio, alle polveri sottili degli scavi per il *tunnel* geognostico del cantiere TAV di Chiomonte, nella ormai distrutta Val Clarea. Clarea. Nonostante tutti abbiano continuato a smentire dati ambientali preoccupanti, come l'allora ministro dei trasporti Maurizio Lupi nell'aprile 2014, durante la discussione sulla ratifica al Senato dell'Accordo tra Italia e Francia, per dare il via libera definitivo, io ho evidenziato la pericolosità dello scavo in Val Susa, sulla base dei dati dell'ARPA di Ivrea e del Politecnico di Torino, che non lasciavano dubbi in merito ai valori allarmanti di uranio e amianto. Avevo chiesto personalmente l'acquisizione di questi dati, per un'attenta valutazione, poiché tutti noi temevamo per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Evidentemente, però, queste sono le umane sorti e progressive, che con l'alta velocità travolgono la vita delle persone e vanno contro natura. Senza contare, poi, il fiume di denaro pubblico. Nelle nostre proposte e valutazioni critiche al DEF 2016, noi avevamo prospettato la possibilità di recuperare circa sei miliardi di euro, rinunciando agli inutili e costosi F35 e alla TAV Torino-Lione. Nessun ascolto, però, ed eccoci oggi a ratificare i lavori definitivi della sezione transfrontaliera. Il nostro contributo, a questo punto, non poteva che rifarsi agli emendamenti, che abbiamo rafforzato con alcune condizioni tassative. Abbiamo chiesto l'integrale attuazione della normativa italiana di contrasto al fenomeno capillare della penetrazione nelle opere pubbliche della criminalità organizzata; che siano preventivamente e precisamente verificate le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati, dalla costituzione di TAV SpA sino alla data di entrata in vigore di questa legge; che sia preventivamente assicurato che il sistema di integrazione della rete garantisca la piena interoperatività e cooperazione fra ferrovie a livello nazionale ed europeo; che siano acclarati i costi complessivi del progetto, individuando quelli sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato per la progettazione, la gestione delle relazioni contrattuali e per altre opere strettamente correlate al progetto. Abbiamo anche posto la condizione che venga istituito un tavolo tecnico cui partecipino tutti i soggetti istituzionali coinvolti e le comunità locali interessate, al fine di verificare se sussistano le condizioni per l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte in comune.

più volte espresso dagli enti locali e dai cittadini, tentando una spregiudicata criminalizzazione di cittadini, intellettuali e artisti che contrastano questo assurdo e diseconomico progetto. Noi ribadiamo che in questa complessa vicenda la concertazione resta un passo fondamentale per arrivare a politiche concrete di tutela dell'equilibrio idrogeologico e paesaggistico dell'area. Sul mancato confronto con gli enti locali e il mondo associativo abbiamo più volte chiesto al Governo di rispondere, in particolare sulla sostenibilità ambientale ed economica dell'intero progetto e sulla necessità di vigilare sulle convenzioni e sugli appalti per la realizzazione dei Faccio un ultimo appello alla ragionevolezza. A me sembra che, a differenza che nel nostro Paese, in Francia, anche se i nostri *media* non ne danno assolutamente contezza e informazione - come su molti altri temi importanti

al parere contrario espresso già due volte dalla Corte dei conti francese, secondo la quale un'eventuale decisione dello Stato di proseguire con questo progetto sarebbe estremamente preoccupante per l'equilibrio futuro delle finanze pubbliche francesi.

non vi è l'attenzione dovuta, non solo alle questioni ambientali, ma al saccheggio delle ultime poche risorse a disposizione del nostro Stato.

di conseguire quei risparmi e quelle ulteriori capacità di trasporto, e si confermano in maniera veramente testarda

già cominciato a far sentire i suoi primi segni drammatici. oggi siamo chiamati a votare il disegno di legge che reca l'autorizzazione alla ratifica ed alla esecuzione di ben tre atti (Accordo, protocollo addizionale e regolamento), nonché dei relativi tre allegati, concernenti l'avvio dei lavori della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Va detto in premessa che il primo Accordo tra Italia e Francia per la costruzione di questo tunnel ferroviario risale al 29 gennaio 2001: sono passati ben quindici anni e stiamo ancora qui a discutere di un tunnel la cui necessità è già stata superata nei fatti. Se sono stati necessari quindici anni per l'inizio dei lavori, quando saranno mai terminati? Visto che amate i pronostici e le lotterie, credo che questi atti servano per implementare il mondo delle scommesse. Come dicevo, sono tre atti fondamentali, formalmente lacunosi, pieni di incongruenze, come è stato ampiamente sottolineato nella discussione generale e dalla questione pregiudiziale. Tra le discrepanze vorrei stigmatizzare il fatto che, per esempio, nell'Accordo viene prevista la possibilità di apportare modifiche nella parte che disciplina la commissione dei contratti, composta da 12 membri, con scambi di lettere - speriamo non con i piccioni - tra le medesime parti. In questo modo si permette che gli eventuali emendamenti proposti sfuggano alla valutazione ed alla successiva ratifica parlamentare. Ricordo che le parti modificabili attraverso scambi di lettere risultano interessare ambiti rilevanti e piuttosto delicati. Un altro elemento di forte criticità dell'Accordo è il trasferimento al promotore pubblico del ruolo di gestore di infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane. sono molto perplesso del fatto che i due rappresentanti dei Governi italiano e francese abbiano firmato l'Accordo riportando la data sbagliata, ovvero retrofissata di un anno. Se non si è capaci di scrivere una data, figuriamoci come si interviene sui contenuti di un Accordo che sono davvero molto complessi. Il secondo atto, il protocollo, prevede all'articolo 2, comma 1, che le parti fissino la stima del costo dell'opera in 8.300 milioni Detto costo sarebbe dovuto essere certificato da una società terza, come stabilito dall'accordo del 2012, ma nel protocollo non ci sono riferimenti alla certificazione di un terzo esterno. Inoltre il costo dovrebbe essere attualizzato, raggiungendo la cifra di 9,69 miliardi Per aggiornare il costo si usa un indice le cui modalità di calcolo sono stabilite nel protocollo stesso, ma il dato interessante è che il protocollo precisa dettagliatamente per il lato francese di spesa il relativo indice di riferimento mentre per i costi del lato italiano si utilizzano generiche ed ambigue indicazioni. Ribadisco ulteriormente che il costo è una stima, quindi non è certo. Inoltre nella certificazione prodotta il 3 maggio 2016 si sottolinea come non sarà possibile perfezionare la stima attuale del costo in base alla soluzione prescelta. Va aggiunto poi che il *grant agreement* stipulato il 25 novembre 2015 assegna un contributo di 814 milioni di euro a fronte di spese programmate di 1915 milioni di euro da realizzarsi entro il 31 dicembre del 2019. Pertanto, allo stato attuale, non vi sono documenti che attestino ulteriori futuri stanziamenti dell'Unione europea. Interessante poi notare nell'articolo 3 l'impegno per prevenire ogni rischio o tentativo di infiltrazione mafiosa, delegando ad una commissione intergovernativa l'incarico di elaborare un regolamento dei contratti estremamente rigoroso. Questo articolo 3 è un capolavoro in quanto, con modalità del tutto singolari quanto improprie, sia l'Accordo che il protocollo producono effetti giuridici internazionali, ossia l'elaborazione di un regolamento dei contratti, prima ancora che i predetti atti siano ratificati e vigenti nell'ordinamento italiano; con ciò facendo si consente che il Parlamento esamini un atto, il regolamento, prima ancora che le fonti del medesimo atto vengano ratificate. Il regolamento si compone di 15 articoli e ben due allegati e ha come oggetto la definizione delle regole applicabili. Al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa, viene costituita una struttura binazionale con due prefetti (uno italiano ed uno francese) che dovranno valutare i titoli delle ditte sulla scorta della *white list* italiana. Abbiamo visto quanto sia complicata la gestione delle *white list* anche in Italia con tutte le nostre banche dati, figuriamoci quando dovremo confrontarci con ditte che hanno sede all'estero, in tutta Europa. Quindi sarà matematico che la *white list* avrà un peso veramente molto ridotto. Diciamo subito che la trasparenza non è una priorità, visto che il direttore generale di TELT (tunnel euralpin Lyon Turin), cioè il soggetto promotore del TAV, è stato rinviato a giudizio per omissione di atti d'ufficio, per non aver reso pubblici gli atti dell'Osservatorio. Speriamo poi che la struttura binazionale sia migliore rispetto a quella di Expo; dopo tanti tavoli tecnici e controlli si scopre che i padiglioni cinese e dell'Ecuador sono stati costruiti da ditte risultate pulite, ma di fatto, come risultato dalle ultime intercettazioni, infiltrate dalla 'ndrangheta. Da ultimo dobbiamo ricordare i dubbi espressi il 10 giugno 2016 dal presidente della Corte dei conti francese, evidenziando come l'Agenzia francese per il finanziamento delle infrastrutture abbia un *budget* ampiamente fuori portata rispetto al costo di questa opera.

Vorrei ricordare solo che saranno movimentati 20 milioni di metri cubi di roccia con concentrazioni di amianto del 1 per cento (a tal fine sappiamo che si sta cambiando il meccanismo regolamentare di questi inerti e si sta alzando la soglia per poterli considerare materiali non pericolosi), 7 milioni di metri cubi di calcestruzzo e un milione di tonnellate di acciaio. Per non parlare poi dell'indebitamento che dovranno pagare le future generazioni, in quanto questa struttura, com'è stato ampiamente dimostrato, non si paga con l'uso, pertanto senza alcun tipo di utilità per il trasporto merci e per il trasferimento modale. trasferimento modale. Gli ingegneri hanno scritto un bellissimo libro sulle ragioni del no, suona bene questo termine; 150 ragioni che smontano punto per punto quanto hanno raccontato su questa inutile e costosa opera, che nessuno ha poi contestato. La cosa che ritengo davvero fondamentale è che sia ben chiaro chi vuole questo tunnel: chi firma gli atti abbia un nome e cognome, perché il tempo passa e quando tutti avranno la matematica evidenza delle nefandezze perpetuate, il responsabile dei fatti dovrà essere certo, non potrà nascondersi nell'anonimato, non potrà dire di aver firmato atti a sua insaputa, che i conti erano sbagliati, che i fatti potevano essere letti in modo diverso. Oggi i giovani valsusini sanno e capiscono: Internet ha la memoria lunga, chiederanno spiegazioni, e voi dovrete dargli una risposta. Non vorrei allora essere nei vostri panni. Detto questo, annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

possano beneficiare di una ripresa economica per la quale bisogna assolutamente impegnarsi. La ripresa è legata anche alla realizzazione di grandi infrastrutture e di investimenti produttivi come questo e non, viceversa, a quello che troppo spesso fa questo Governo, indebitando il Paese per aumentare sensibilmente la spesa corrente. Vorrei, poi, ricordare che questa infrastruttura beneficia di un contributo dell'Europa. Ci lamentiamo che l'Europa fa poco - ed è vero e lo diciamo con

un po' folkloristiche, tipo togliere le bandiere europee o altro, che il Governo sta realizzando in questi giorni. Signor Presidente, per queste motivazioni, che ho cercato di sintetizzare, Forza Italia voterà convintamente a favore di questa ratifica. Signor Presidente, con la ratifica di questo Accordo tra Italia e Francia si arriva a conclusione di un lungo percorso - forse troppo lungo per la realizzazione di un'opera, non solo definita strategica dal Governo italiano e dal Governo francese, ma voluta fortemente, come dimostrano l'interesse, l'attesa e il contribuito economico che è stato messo in campo, anche dall'Unione europea. Si sente spesso parlare di ambiente. Da più parti ci si riferisce a questa linea ferroviaria come a un'opera che danneggia l'ambiente. La nuova linea Torino-Lione è invece un'infrastruttura che salvaguarda l'ambiente. Voglio ricordare che ogni anno, sulle Alpi, nella parte italofrancese, 2,5 milioni di mezzi pesanti attraversano le nostre strade, con un impatto ambientale che credo non sia necessario ricordare. L'Europa - quella che ci piace, quella che lavora anche attraverso le reti di comunicazione a costruire una vera sensibilità europea e non solo l'Europa dell'austerità

Questa strategia riguarda anche gli impegni presi dall'Europa - se ne è parlato in quest'Aula nelle scorse settimane - per la riduzione dei gas serra. L'obiettivo che ci si pone e che sarà realizzato con l'entrata in funzione di questa nuova linea sarà di togliere un milione di mezzi pesanti dalle strade italiane e francesi all'altezza delle nostre Alpi. Alpi. La linea storica di cui molto - forse troppo - si parla fu voluta, devo dire con grandissima lungimiranza, da Camillo Benso di Cavour: è un tunnel ferroviario del 1871 che ha dato la possibilità di sviluppare

con tutti gli sforzi di ammodernamento possibili, è un'infrastruttura che non ha la possibilità di svolgere quella funzione di togliere i camion dalla strada per metterli sulla ferrovia. Ricordiamoci sempre che l'interscambio tra i Paesi dell'area (Francia, Spagna e Inghilterra), cioè quelli che saranno interessati dall'utilizzo di queste infrastrutture, è di 40 milioni di tonnellate l'anno e vale 130 miliardi. Questo spiega bene le ragioni per le quali l'Europa, per una volta non dimenticando il libro bianco di Jacques Delors, che parlava delle reti infrastrutturali come della vera realizzazione dell'Europa, come delle arterie attraverso cui far scorrere davvero i rapporti all'interno dell'Europa, ha messo un contributo rilevante, pari al 40 per cento. Questa è una delle opere europee maggiormente cofinanziate. Permettetemi di dire un'ultima cosa. Si parla spesso delle infiltrazioni nelle grandi opere e si cita a sproposito quello che avviene sul terzo valico. Vorrei ricordare che quest'opera non la realizziamo con il contraente generale, né con quei meccanismi che quest'Assemblea, il Partito Democratico e molte forze politiche con il nuovo codice degli appalti hanno deciso di

terzo (perché la Francia è un Paese terzo rispetto a noi). Questo è un rilevantissimo passo in avanti nelle relazioni europee e nella comprensione, da parte degli altri Paesi del fenomeno delle infiltrazioni e della criminalità, che come sappiamo travalica i confini. È anche un grandissimo successo del Governo italiano e di tutti quelli che hanno creduto e che credono nella possibilità di realizzare grandi opere tenendo fuori la criminalità organizzata i mafiosi e soprattutto ponendo grandissima attenzione al raggiungimento degli obiettivi nei costi stabiliti. Questo Accordo è la certificazione finale di tutto ciò. Oggi è una giornata molto importante, perché chiudiamo il processo di approvazione e

con il raggiungimento di un obiettivo: quello di dire oggi che ci sarà un'opera pubblica, una grande opera pubblica internazionale, i cui costi sono codificati. Non dovremo più rincorrere, come spesso è avvenuto in questi anni, l'aumento inutile dei costi a danno dei soldi dei contribuenti. I cittadini italiani oggi sanno che quell'opera ha un costo definito, controlli certi e una normativa che impedirà alla criminalità organizzata di attraversare il confine e di utilizzare norme più favorevoli, perché le norme antimafia sono quelle italiane e saranno norme che garantiranno la trasparenza. Per questa ragione, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, onorevole Marianna Madia, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: ripresa della contrattazione nel pubblico impiego; riforma della disciplina della dirigenza pubblica.

che è avvenuto quello che noi dell'Italia dei Valori avevamo preannunciato quando ho parlato della mozione che abbiamo presentato in Senato per risolvere il problema dell'epatite C.

visto che attualmente, in ragione dei costi, ci possiamo permettere di trattare solo i casi più gravi. Abbiamo anche visto che esiste un commercio parallelo

Che per gli alti costi di un farmaco ci venga impedito in Italia di poter trattare le persone più giovani, che sono poi quelle che trasmettono la malattia, lo ritengo un assurdo e una discriminazione che